Dopo l’approvazione del calendario, la seduta sarà tolta per consentire alla Commissione finanze di terminare l’esame del decreto-legge recante misure a favore di investitori in banche in liquidazione. La discussione in Assemblea del provvedimento, fino alla sua conclusione, avrà luogo nella seduta unica di domani per la quale non è previsto orario di chiusura. La Presidenza potrà disporre sospensioni in relazione all’andamento dei lavori. Lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni è rinviato alla seduta pomeridiana di giovedì 23 giugno. La prossima settimana l’Aula non terrà seduta in vista del secondo turno delle elezioni amministrative. L’Assemblea tornerà quindi a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 21 giugno. Il calendario prevede le mozioni sulle concessioni demaniali marittime e contro la corruzione negli appalti; ratifiche di accordi internazionali; il disegno di legge in materia di mandati degli organi del CONI; il decreto-legge proroga missioni internazionali e il collegato sulla semplificazione del settore agricolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. lunedì 27 giugno, alle ore 11, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà le proprie comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno.

quella antecedente al turno di ballottaggio, per un motivo fondamentale: le persone coinvolte nel turno di ballottaggio stanno lavorando, lo stanno facendo anche in questo momento e non credo che i nostri colleghi parlamentari saranno attivi la prossima settimana. È già successo la scorsa settimana e lo stesso avverrà alla Camera, quindi siamo contrari a questo calendario. BELLOT

Banca d’Italia e il suo Governatore dovrebbero operare. Si tratta di una mozione che abbiamo chiesto già ai primi di gennaio di calendarizzare e di cui continuiamo a chiedere la calendarizzazione. Chiediamo che trasparenza e giustizia siano fatte proprio andando ad incidere su chi ha operato in maniera a nostro avviso non corretta e comunque,

Presidente, è un argomento che si trascina ormai da troppo tempo. Noi chiediamo che venga

si stabilirebbero delle priorità di esame in vista delle decisioni assunte per quanto riguarda il calendario. Un po’ mi avete preso in parola, nel senso che abbiamo fatto una programmazione fino alla

sono passati quasi due mesi dall’approvazione della mozione che impegnava il Governo a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze.

scusi se mi permetto di puntualizzare questo aspetto ma, essendo lei la figura più autorevole in questo consesso,

seria riflessione sul dare dignità a noi senatori, a noi parlamentari che svolgiamo questo ruolo e soprattutto ai cittadini che rappresentiamo. Signor Presidente, ancora una volta, cortesemente, si impegni affinché questo avvenga. Lo faccia,

Signor Presi- dente, intervengo brevemente per ricordare che esattamente trentasei anni fa, l’8 giugno del 1980, moriva in seguito ad un incidente stradale Bruno Salvadori. Nato ad Aosta nel 1942, Bruno Salvadori si dimostrò sin da subito sensibile alla causa autonomista e federalista, aderendo all’Union Valdôtaine e dimostrando spiccate doti di comunicatore e di giornalista. La militanza politica attiva lo portò a ricoprire il ruolo di consigliere regionale e direttore del giornale del movimento, «Le Peuple Valdôtain», ma uno dei suoi maggiori fu quello di aver portato fuori dalla Valle d’Aosta l’idea di federalismo, con l’intento di far conoscere il più possibile questo modello di organizzazione dello Stato, che da sempre è il punto di riferimento del pensiero autonomista.

mentre stavo partendo, mi è stata recapitata una lettera che ritengo necessario trasformare in interrogazione, per capire se il contenuto della stessa trovi corrispondenza o meno, perché, signor Presidente, come potrà apprendere dal contenuto della stessa, contiene profili quantomeno inquietanti. «Sono un lavoratore della Sogepu. In questi giorni c’è la campagna elettorale e i lavoratori interinali della Sogepu sono stati riuniti e si sono presentati il presidente Cristian Goracci insieme a Luca Secondi, assessore all’ambiente. Ai lavoratori hanno detto che sarebbero stati assunti dopo le elezioni, ma dovevano dare il voto all’assessore, loro e le loro famiglie. Abbiamo avvertito i sindacati che hanno chiamato il Comune, ma nessuno ha detto niente. Li hanno avvertiti che se non fosse stato eletto Luca Secondi, non ci sarebbero state le assunzioni. Verificate se quello che dico è vero; chiedetelo pure ai lavoratori e ai sindacati della Sogepu per vedere se è vero. Questa gente non deve essere votata, perché specula sulla povera gente con i nostri soldi. Promettono un posto di lavoro per i voti. Vi chiediamo di controllare, ma fate qualcosa». Signor Presidente, ritengo che questo fatto sia necessariamente da verificare. Anticipo quindi un’interrogazione al Ministro dell’interno,

ma due settimane fa ho chiesto che venisse data risposta all’interrogazione 3-02831 riguardante l’intento di Poste Italiane di procedere il prossimo 13 giugno (cioè fra cinque giorni) ad iniziare l’attività di recapito a giorni alterni tutta la corrispondenza nelle zone disagiate o difficilmente raggiungibili. Il recapito della posta a giorni alterni è in funzione in altri Paesi del mondo, anche avanzati, anche in alcuni territori degli Stati Uniti d’America. Ma una cosa deve essere chiara: che la normativa di tutto ciò che significa notifiche e di tutto ciò che riguarda i diritti dei cittadini deve essere adeguata. Siccome le Poste svolgono un servizio universale, a giorni alterni, che sia così per tutta Italia, adeguando la relativa normativa per tutto ciò che riguarda il servizio di notifiche e quant’altro. Ciò che non è tollerabile

pertanto al sottosegretario Pizzetti di interessarsi di nuovo, visto che l’ha fatto la scorsa volta con estrema gentilezza ma non abbiamo ottenuto il risultato, e di avere una risposta del Governo

dello Stato un servizio essenziale ed importante, che prevede che esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Siccome a mio avviso questo è inaccettabile, attendo la risposta perché il Governo confermi,

Bruno Salvadori è stato un grande valdostano e un grande ispiratore della trasformazione forse più importante che c’è stata in questo Paese.

Chi ben conosceva l’autonomia, poteva capire che non bastava avere dallo Stato deleghe, ma bisognava avere competenze primarie: siamo noi che riconosciamo che lo Stato ci rappresenta, non è lo Stato che

Noi riconosciamo Salvadori come un padre putativo della Lega, così come lo fu il grande professor Miglio, e ricordiamo che la terna Miglio-Bossi-Salvadori

la prima riforma in senso federalista dello Stato. Tanto ancora c’è da fare, ma crediamo che questo nostro Paese dovrebbe ricordare e

n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (2362 ) La seduta è tolta